non solo noi, ma tutta l'opinione pubblica è rimasta profondamente colpita dalla campagna pubblicitaria promossa dalla ministra Lorenzin sul cosiddetto Fertility day*,* in cui emerge un'immagine - peraltro quasi minacciosa - della donna con la clessidra, che richiama a nostro avviso l'antica idea della donna ridotta solo a corpo e natura e obbligata a fare figli. Si tratta, quindi, di un messaggio a nostro avviso assolutamente regressivo e di forte impronta ideologica.

Il tema della denatalità, al contrario dell'impronta ideologica e aggressiva che si è voluta dare alla campagna di comunicazione, è molto serio. molto serio. I dati dell'ISTAT evidenziano come i nuovi nati siano in costante diminuzione: nel 2015 le nascite sono state 488.000 (-15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La decisione di mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come documenta ormai l'aumento dell'età media delle madri al parto. parto. Noi riteniamo che affrontare questo problema così serio da parte del Governo e del Ministero a colpi di pedagogia autoritaria sia assolutamente fuorviante fuorviante e inefficace, perché rinunciare o rimandare la scelta di fare un figlio sta dentro una complessa serie di ragioni che riguardano non solo la soggettività (in cui ovviamente si intrecciano sessualità, amore, futuro, libertà, relazione tra i sessi e fiducia nel futuro) e che non possono essere né semplificate con richiami volontaristici né tantomeno ricondotte solo a parametri sociali ed economicisti. La bassa crescita o la decrescita demografica è, in primo luogo, un problema che deve essere affrontato in una dimensione globale. Un piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve muovere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e del diritto alla salute riproduttiva e soprattutto dal promuovere robuste politiche attive e strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scelte di vita che creino le condizioni di sostegno alla scelta di fare figli. un nuovo sistema di *welfare* e in esso più servizi socio-educativi: riconoscimento sociale della cura, sostegno al reddito, congedi parentali incentivanti per gli uomini, più lavoro femminile organizzato per poter accudire le relazioni umane. Molte realtà europee dimostrano che c'è un rapporto diretto tra accesso femminile al lavoro, natalità e benessere generale. L'Italia si conferma invece uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, e questo condiziona fortemente la stessa possibilità di determinare il proprio progetto di vita. I dati del Rapporto Italia 2015 dell'Eurispes hanno evidenziato l'incidenza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nella crescita del numero di chi non si sente in grado di dare garanzie alla propria famiglia con il proprio lavoro. Queste sono le questioni vere

anche di un messaggio razzista. Pertanto, nella nostra mozione chiediamo con molta decisione non solo di cancellare definitivamente la campagna, ma di assumere iniziative per prevedere che il 22 settembre diventi davvero una giornata di formazione e informazione sul diritto alla salute riproduttiva per la prevenzione della fertilità; di affermare il principio della libertà nelle scelte procreative; di investire risorse finalizzate davvero a un piano di prevenzione della sterilità; di assumere iniziative per garantire l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita in tutto il territorio nazionale, promuovendo la conoscenza e la pratica

visto che entriamo nella sessione di bilancio, di assumere iniziative per chiare scelte di politica economica, sociali e strutturali, volte a sostenere l'autonomia delle persone, rimuovendo gli ostacoli sociali che possano condizionare il desiderio il desiderio della maternità. Chiediamo, inoltre, un piano straordinario di promozione e sostegno al lavoro femminile con incentivi e modalità organizzative basate sui nuovi rapporti tra produzione e riproduzione, nonché il riconoscimento sociale e la valorizzazione del lavoro di cura anche con lo sviluppo di infrastrutture sociali di stampo europeo e di assumere efficaci iniziative anche nell'ambito dell'Unione europea volte a prevedere l'esclusione del rispetto del Patto di stabilità per le spese relative ai servizi sociali e al *welfare*. In ultimo, ma non per importanza, chiediamo di assumere iniziative per riconoscere il tempo dedicato alle attività di cura ai fini pensionistici (con il riconoscimento dei contributi figurativi legati al numero di figli ed eventuali altri impegni di cura per altre persone anziane in famiglia, nonché con il riconoscimento di integrazioni contributive per i periodi di lavoro *part-time* per ragioni di cura e possibilità di anticipo della pensione per necessità di accudimento di persone non autosufficienti), nel quadro di una revisione del sistema pensionistico

per le donne lavoratrici, con particolare riguardo alle piccole e micro imprese, sulle quali i costi incidono in misura proporzionalmente maggiore.**

definendola una primipara attempata che sta svolgendo un ruolo prevalentemente maschile, avendo in maniera narcisistica percorso un profilo di studi che l'ha, in maniera egoistica, tolta da quella che era la sua reale funzione, ossia di mettere al mondo dei figli per garantire il *welfare*, lei pensa che potrebbe sentirsi colpita da questo tipo di affermazione? Perché la campagna pubblicitaria con la quale il Ministro voleva porre l'attenzione sul problema serio della denatalità è solamente la punta dell'*iceberg* di un Piano nazionale per la fertilità che,

«La conferma del modello della famiglia unicellulare, con il primo figlio procreato da primipare attempate…». attempate sono donne che, probabilmente, prima di mettere al mondo un figlio, hanno dovuto studiare, lavorare, crearsi una posizione, trovare una casa, dare dignità alla propria persona e dare la possibilità al figlio che mettevano al mondo di avere, quantomeno, la sicurezza che la mattina ci fosse una colazione e la del senatore Campanella)*. Queste sono le primipare attempate. E queste stesse primipare si ritrovano in una società che ha dovuto scortare le donne fuori casa, aprendo loro le porte del mondo del lavoro, sospingendole, però, verso ruoli maschili.

fertilità, i ruoli che la donna deve ricoprire all'interno della società per garantire il *welfare*. Perché questo dice la Lorenzin. Dal momento che le donne non fanno figli, noi non riusciamo a garantire il *welfare*. Io vorrei dire alla Lorenzin che, se fosse garantito un *welfare*, probabilmente le donne farebbero dei figli. Ma una donna normale non ha la possibilità, di ricevere uno stipendio di quasi 20.000 euro e non ha la possibilità, come ha invece il Ministro, di godere di un'assicurazione che le ha consentito, probabilmente, di non dover fare la richiesta

sanitario le è garantito dall'assicurazione privata che la Camera mette a disposizione. Perché voi non sapete? Perché il Ministro si permette di scrivere che l'istruzione delle donne è uno dei motivi che ha portato alla scelta egoistica di non fare figli? Ma

una notevole fatica a conciliare, la mattina quando ti alzi, la colazione ai tuoi figli, con il portarli a scuola, andare a lavorare, tornare a casa, fare la spesa, ripulire la casa? Perché lo fai? Ma stai a casa! Non studiare! vent'anni fai un figlio, quando ancora le tue ovaie sono in grado di procreare, tanto tuo marito può farlo fino a settant'anni. Fuori dalla campagna propagandistica vergognosa, che vedeva la donna con la clessidra in mano e in attesa della cicogna, e fuori dalla seconda campagna vergognosa, che addirittura vedeva la donna sana se è bionda e bianca, e malata se è di colore differente o eventualmente sta fumando una sigaretta, c'è veramente uno scollamento dalla realtà. Se la Lorenzin vuole veramente fare qualcosa per le donne, lasci il ruolo di Ministro della salute a qualcuna che forse è più in grado di lei di capire cos'è una donna.

non mi dilungherò sul testo della mozione; voglio solo brevemente puntualizzare alcune semplici considerazioni che l'hanno ispirata. La campagna ideata e promossa dal Ministero della salute in occasione dell'evento denominato Fertility day ha provocato un'ondata di malcontento in un'ampia parte dei cittadini, soprattutto donne, che forse negli intenti dovevano essere le destinatarie principali di questa iniziativa. Inizierei dall'opportunità dell'iniziativa in sé: una giornata dedicata alla fertilità, quindi alla procreazione, promossa da un Governo che non ha saputo prendere alcuna altra iniziativa a sostegno della maternità e della famiglia più in generale. Nessun risultato serio in questi due anni di Governo in merito alla diminuzione della disoccupazione giovanile o alla tutela delle lavoratrici madri. Nessuna azione o iniziativa efficace per affrontare il problema casa, il problema degli asili nido; per non parlare poi del taglio delle prestazioni sanitarie legate soprattutto alla prevenzione e alla diagnosi precoce, per le quali gli italiani devono ormai ricorrere alle strutture private. Il *mantra* è sempre lo stesso: non ci sono le risorse. Ed è proprio per questo che chiediamo al Governo di impegnarsi a verificare e rendere pubblico il costo che il Ministero ha sostenuto per le due campagne ritirate. Inoltre, al fine di una definitiva chiarezza relativamente ai fatti avvenuti, chiediamo che il Governo si impegni a chiarire a rendere pubblici il processo decisionale vigente presso il Ministero della salute e la regolamentazione degli istituti della delega e delle autorizzazioni. Infine, nel rispetto dei nostri cittadini, soprattutto di quelli che, non godendo di agiatezza economica, sono più vulnerabili, chiediamo che il Governo, verificate le responsabilità in merito alla vicenda delle campagne promozionali ritirate, si impegni a percorrere ogni possibile azione di rivalsa per riportare il denaro pubblico così inutilmente speso nella disponibilità del Ministero, con l'auspicio di vederlo poi destinato ad azioni o iniziative maggiormente coerenti con le ormai impellenti necessità delle persone. Ha facoltà di parlare la senatrice De Biasi per illustrare la mozione n. 644. *(PD)*. Signor Presidente, non v'è dubbio che una campagna di comunicazione, assai scadente peraltro dal punto di vista comunicativo e professionale, prima ancora che nei contenuti sanitari, ha modificato la percezione dell'opinione pubblica e dello stesso Parlamento sulle finalità del progetto sulla fertilità, cioè del Piano nazionale per la fertilità, che come sappiamo appartiene al Ministero nella sua autonomia e che, come nel caso

della doppia campagna comunicativa ha ulteriormente oscurato contenuti che, viceversa, vanno segnalati. Innanzitutto, il primo elemento è che non bisogna confondere il tema della fertilità, ammesso che si possa chiamare in questo modo, con quello della natalità. Credo che la parola «fertilità» si possa lasciare a una parte della letteratura scientifica che viceversa il termine opportuno sia «salute riproduttiva» delle donne e degli uomini. Sappiamo bene ciò che questo comporta anche relativamente alla legislazione italiana, in parte ancora da correggere - penso alla legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che pregherei di non chiamare più sulla fecondazione assistita perché si tratta di procreazione medicalmente assistita in particolare perché vanno ottemperate le sentenze della Corte costituzionale. C'è un tema di carattere sanitario che riguarda la salute

per lo sviluppo della consapevolezza della propria sessualità. Vorremmo che in questo Paese ci fosse una contraccezione seria una contraccezione seria che non intervenga solo sul corpo delle donne e che non sia esclusivamente riparativa, collocandosi all'interno di una strategia di prevenzione. Da questo punto di vista, chiediamo che si torni indietro dalla decisione

efficace e, penso, anche diffusa e gratuita. Noi chiediamo che si torni indietro su questo punto, come chiediamo che del Fertility day si possa parlare con la lingua italiana e si chiami «Giornata della salute riproduttiva»,

denatalità. Sovrapporre i due piani è un'operazione molto scorretta, perché non possiamo essere così sommari e pensare che vi sia un automatismo tra condizioni economiche e possibilità di fare figli. C'è una relazione indubbia, ma non si ferma lì; lo dobbiamo alle persone sterili, alla mancata ricerca sulle cause della sterilità e particolarmente di quella maschile, su cui non si dice mai niente perché si parla sempre e solo delle donne.

Vorrei però tornare al punto di carattere sanitario e socio sanitario, su cui ci siamo esercitati a lungo, anche nel dibattito sulla riforma costituzionale. C'è un servizio che si chiama consultorio, che è stato approvato con una legge del 1975, Questo servizio dovrebbe servire esattamente a essere un momento di intercettazione del bisogno delle persone sulla propria salute riproduttiva. È un servizio

c'è bisogno di riforme forti, a partire dalla legge n. 40 del 2004, ma c'è soprattutto bisogno - lo devo dire anche per la storia delle donne di questo Paese - di un piano più serio di quanto non sia stato fatto finora sulla vita e sulla salute riproduttiva delle donne, dall'adolescenza - con i vaccini contro il papilloma *virus* - fino al parto e al dopo parto. Sulla scelta e libertà consapevole di essere o non essere madre ancora oggi siamo

una grande occasione è andata perduta: quella di poter discutere, o almeno aprire un importante dibattito culturale su un tema che riguarda il nostro Paese come tutti i Paesi sviluppati e il fronte occidentale nel suo complesso. L'istituzione di una giornata nazionale dedicata al tema che, come ha già detto la senatrice De Biasi, forse era meglio chiamare in modo diverso da Fertility day, poteva rappresentare un'occasione per richiamare l'attenzione su come la nostra società si va componendo o scomponendo e su dove sta andando. Si trattava di mettere semplicemente a fuoco, anche se con grande enfasi, il pericolo della denatalità, la bellezza della maternità e della paternità, il rischio delle malattie che impediscono di diventare genitori,

hanno completamente deviato l'attenzione dal vero tema in questione e hanno fornito degli splendidi *assist* alla satira e al *web*. Ma non c'è da ridere. Non c'è da ridere quando l'immagine che ha voluto rappresentare questa campagna ha dipinto le donne come yogurt in scadenza. Inutile ribadire che è per noi sacrosanta una politica che si occupi della salute delle donne, dalla nascita alla procreazione fino alla menopausa, come lo sarebbe una educazione sessuale nelle scuole, che aiuti a crescere ambo i sessi nel rispetto reciproco, nell'amore e nella conoscenza, cui oggi purtroppo gli gli adolescenti giungono più spesso attraverso altre modalità, tutte legate alla rete, e talvolta con nefaste conseguenze. accusano le italiane di fare troppo pochi bambini. Ma vogliamo ricordare che da noi gli asili nido sono un bene raro e costoso? Per non parlare della piaga di una disoccupazione femminile della quale sembriamo non liberarci mai? Potremmo andare avanti con statistiche, che non esauriscono però l'indignazione provocata da questa campagna. Bisognerebbe leggere tutto il documento per arrabbiarsi definitivamente, come ha fatto la senatrice Taverna prima, il punto dirimente è racchiuso in alcune frasi di questo tipo: «Cosa fare, dunque, di fronte a una società che ha scortato le donne fuori di casa, aprendo loro le porte nel mondo del lavoro sospingendole, però, verso ruoli maschili, che hanno comportato anche anche un allontanamento dal desiderio stesso di maternità?». Sottosegretario De Filippo, lei, oltre ad essere così squisito da essere presente stamane, dovrebbe raccontare al suo Ministro che le parlamentari di quest'Assemblea stanno mettendo in evidenza come il suo ruolo sia stato pesantemente inficiato da un approccio che non so se sia farina del suo sacco. Certo, probabilmente, è farina del sacco di chi, selezionato malamente, ha riversato in questa campagna tutto il suo banale maschilismo.

le donne romane quando il buon Augusto, per incoraggiare la fertilità (anche all'epoca c'era la necessità di un Fertility day) impose a tutte, salvo alle prostitute, di sposarsi, punendo chi non poteva avere figli. Per protesta, le cittadine romane andarono in massa a iscriversi nelle liste delle prostitute, per sbeffeggiare l'imperatore.

Ci dispiace molto, come donne, sapere di avere un Ministro donna, peraltro madre da poco tempo (anche lei forse una puerpera un po'

non arrivano, soprattutto nei mesi più delicati in cui una donna affronta tutto questo, quando proprio quel sistema sanitario che dovrebbe proteggerla, tutelarla, darle una corsia preferenziale e mostrare un volto del tutto diverso da quello che caratterizza il suo modello organizzativo, la

educazione possa aiutarci a prevenire una distorsione del tema della maternità, quale può essere considerato l'aborto. Tanta strada è stata fatta dalle donne che ci hanno preceduto. In questo Parlamento oggi si celebra una censura a un Ministro che ha fatto fare chilometri indietro alla cultura e alla dignità delle donne. Non dovremmo essere noi a chiederle di dimettersi, ma dovrebbe capire da sola che ha dimostrato ampiamente di non poter ricoprire quel ruolo. Abbia la decenza di dimettersi e restituire alle donne italiane il primato di un ruolo, come quello del Ministro della salute, che tante altre donne hanno svolto con impareggiabile

alle attività poste in essere dal ministro Lorenzin. Ciò che più stupisce però è l'intervento della Presidente della Commissione sanità del Senato.

se la critica al ministro Lorenzin parte dal suo interno, credo che anche il Presidente del Consiglio dei ministri e lo stesso Governo dovrebbero cominciare a fare una riflessione seria in ordine alla capacità del Ministro di rappresentare le linee del Governo.

coglie un aspetto che, per la verità, avevo già colto e che trovo di una gravità inaudita:

è un tema che ho attenzionato; forse è sfuggito ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che ne avrebbero dovuto fare una battaglia e forse ne avrebbero avuto anche più titolo di me.

per campagne pubblicitarie del tutto scostumate nei confronti delle italiane, degli italiani Gioca a fare il Ministro e tralascia di considerare che forse, se impegnasse il suo tempo a trattare a trattare con l'America l'acquisto di questo farmaco al pari degli altri Paesi, forse noi vedremmo più cittadini godere di questo beneficio. In Campania - e mi rivolgo

si sente rispondere dal centro che la cura non gli può essere data perché è stato stabilito che chi ha oltre settant'anni deve morire e non deve campare. Io, per la verità, anche se Dio o una una Santa mi dicessero una cosa del genere, probabilmente reagirei violentemente. Se poi me lo dovesse dire una gentile signora

garbate - ma sempre critiche restano - della presidente della Commissione sanità De Biasi. Chiedo pertanto di sottoscrivere la mozione a prima firma della

È iscritto a parlare il senatore Campanella. Al di là delle considerazioni e delle citazioni di norme e situazioni precise, la nostra società non sta bene, i nostri giovani non stanno bene. In genere, quando si sceglie consapevolmente di fare un figlio,

conto di ciò, provare a immaginare un aumento della disponibilità a procreare attraverso una campagna pubblicitaria dà il senso di uno scollamento netto con la realtà.

la spesa per l'assistenza e la sicurezza durante il parto. D'altro canto, la rete di protezione sociale viene meno

Signor Presidente, ringrazio veramente senza problemi le senatrici e i senatori per aver voluto richiamare nuovamente l'attenzione su un tema,

La Giornata nazionale è finalizzata - questi sono gli obiettivi - ad aumentare nella popolazione, soprattutto nei più giovani, la conoscenza della propria salute riproduttiva, fornire strumenti per tutelare la fertilità di uomini e donne attraverso azioni di prevenzione (abbastanza note nel nostro sistema sanitario italiano, anche se difformemente realizzate, e non sistematicamente, come si prevede e si impegna a fare questo piano); la diagnosi precoce e la cura di malattie sessualmente trasmissibili, che possono - come è noto a noi tutti - compromettere il a noi tutti - compromettere il futuro di scelte ontologicamente libere nella vita delle persone, nonché a fornire i giusti elementi di conoscenza sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che

è stato compilato sulla base di valutazioni, che mi sentirei di definire tecniche, scientifiche, da un gruppo ampio di scienziati di orientamento culturale assolutamente vasto, vasto, trasversale, che dovevano sorreggere un'iniziativa del Ministero sottraendolo da un dibattito che in questa materia può essere

In questo senso, anche l'Organizzazione mondiale della sanità, proprio alcune settimane fa, ha adottato una risoluzione, all'interno del Comitato regionale europeo della stessa Organizzazione, con cui i Paesi della regione europea si sono impegnati ad attuare il Piano d'azione si chiama proprio così - per la salute sessuale e riproduttiva nel nostro Continente. In questo contesto e con queste oggettive, e per molti aspetti semplici, finalità, possiamo riassumere e valutare la portata di quella giornata del 22 settembre, e cioè un'occasione per avviare - è stato avviato anche con qualche elemento di

ai mezzi di comunicazione e a coloro che si vogliono occupare correttamente di questa materia in termini di informazione. Il Piano nazionale fissa proprio questo principio - lo vorrei sottolineare perché è stato richiamato nel dibattito - per favorire la natalità. Se da un lato è imprescindibile lo sviluppo di politiche intersettoriali, ovviamente forti, e interistituzionali a sostegno della genitorialità - e nelle mozioni sono state trascritte molte condivisibili

buone pratiche conosciute in alcune parti del nostro Paese, che speriamo si possano diffondere in maniera più consistente e uniforme a livello nazionale. A questo riguardo - e concludo

tutto ciò che è in sintonia con quanto ho voluto velocemente descrivere. Con riguardo invece alle parti che hanno una connotazione di valutazione istituzionale e politica,

sulla mozione n. 645 della senatrice Bonfrisco. Chiederemmo di espungere, nelle premesse, i paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 e 19

Signor Presidente, sarò brevissima. Innanzitutto vorrei ringraziare il sottosegretario De Filippo per la sua gentilezza. svuotare una mozione nei suoi punti fondamentali non è un buon modo per affrontarla o per poterla condividere con il Governo. Mi rendo conto

tuttavia notare le profonde contraddizioni esistenti tra l'azione del Ministro e la mozione della senatrice De Biasi. Vi invito quindi a fare pace almeno tra di voi e - come vi ha già ricordato il senatore Falanga affrontare la questione come va fatto veramente. Aggiungo che le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il messaggio fortemente razzista e penalizzante per le donne italiane, che la seconda campagna diffondeva, sono state affrontate dal ministro Lorenzin sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile della comunicazione del suo Dicastero. Gli importi stanziati per la campagna risultano essere di 113.000 euro e l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata scelta tramite un bando pubblico indetto il 18 dicembre 2015 e chiuso dieci giorni dopo: una rapidità davvero encomiabile in un'attività ministeriale e burocratica che di solito che di solito prende molto più tempo e si muove con maggior lentezza; evidentemente la rapidità serviva a selezionare un'agenzia pubblicitaria che era talmente condivisa dalla struttura e dal Ministro che non poteva che fare bene e invece - come avete visto - ha fatto molto male. Quel danno economico arrecato alla collettività italiana e alle tasse che i cittadini pagano speriamo sia in qualche modo sanato da qualcuno che, sotto la sua responsabilità personale, risponda di un'azione così sbagliata. Il Ministro continuerà a rispondere del ruolo che non riesce a svolgere, che non è capace di svolgere, su questo fronte come su molti altri. Comprendo benissimo la *realpolitik* del sottosegretario De Filippo; a voi lascio la mozione di maggioranza insieme al suo Ministro, mentre a noi dell'opposizione non resta che stigmatizzare ancora una volta l'atteggiamento di un Governo che mette la testa sotto la sabbia e non sa affrontare realmente i problemi.

questa campagna pubblicitaria che doveva portare ad un esito diverso da una semplice mozione. Presidente, in interventi di fine seduta già tre o quattro volte le ho chiesto di

non un controllo di sponsorizzazione di 50.000 euro per la festa di Comunione e Liberazione, di 700.000 di anticipo di stipendio al presidente o all'amministratore delegato di Aifa.

intervenendo sulla salute, sia un dovere di tutti quanti noi e in ciascuna mozione, di maggioranza o minoranza, lo spirito è finalizzato ad andare incontro alla salute dei cittadini. Per questo, responsabilmente, le voteremo tutte. conclusione, mi associo a chi sostiene che il Ministro debba avere il coraggio di venire qui perché, se non lo fa, è bene che non stia nemmeno al Ministero della salute. abbiamo ascoltato le parole del sottogretario De Filippo e comprendiamo le sue difficoltà. Ci ha spiegato l'impegno del Governo sulle politiche sanitarie, ma comprendiamo la pacatezza con cui ha parlato. È chiaro a tutti, infatti, che siamo dinanzi a una vicenda incredibile, a dir poco imbarazzante, per un Paese europeo nel 2016. 2016. Il tema oggi in discussione riguarda la scelta del Governo della campagna sul Fertility day che ha sorpreso tutti. penso anche a molti di coloro che sono al Governo, a partire dal Presidente del Consiglio. Dopo anni di tagli alla sanità pubblica, con milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure, con un *welfare* pubblico assente, il sostegno alla maternità inesistente, tagli senza fine all'istruzione e ai servizi, tutto a vantaggio dei privati, ci siamo ritrovati dinanzi alla campagna pubblicitaria del Fertility

in quale Paese abbia vissuto in questi anni; se fosse rimasta qui, con gli occhi rivolti al Paese reale, si sarebbe accorta che, se in Italia non si fanno figli, è perché il *welfare* pubblico non esiste. Non esistono serie politiche a sostegno della maternità. Non esistono politiche per il lavoro. L'ascensore sociale è fermo e non esiste un Governo che paia voler cambiare rotta rispetto ai regali ai privati, alla progressiva privatizzazione del Sistema sanitario, alle politiche di austerità, ai tagli ai servizi. Se vogliamo parlare della fertilità dal punto di vista sanitario, ci spieghi allora la Ministra i ritardi e le difficoltà di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, dopo lo strazio che è stato fatto della legge n. 40 del 2004, che la destra, della quale lei rimane ancora una illustre esponente, ha votato e rivendica con orgoglio. Parliamo di stili di vita, di progetti educativi, di tante proposte attuabili solo se c'è la volontà di trovare le risorse. Se vogliamo parlare di fertilità dal punto di vista sociale e demografico, affrontiamo allora i problemi che costringono i giovani a rinviare la scelta di fare figli. Se vengo assunta grazie al *jobs act* ma pagata in *voucher*, ovviamente non penserò alla clessidra che scorre, perché ho il problema di come sopravvivere quotidianamente. E se parlare di fertilità vuol dire disegnare la donna come una fattrice in scadenza, allora sarebbe stato meglio stare zitti. Al contrario, sarebbe stato utile e urgente parlare di natalità, di salute riproduttiva, di genitorialità consapevole, di interruzione della gravidanza da garantire nel servizio pubblico, di rifinanziamento dei consultori giovani, di prevenzione e politiche per la contraccezione ma, soprattutto, introdurre, ad esempio, l'ora di educazione sessuale nelle scuole. Eppure, di tutto questo non abbiamo parlato. Ci dispiace dire che è apparsa chiara a tutti i cittadini la totale inadeguatezza della ministra Lorenzin. le nostre convinzioni si sono addirittura rafforzate con la seconda parte della campagna, che definire vergognosa è poco; le buone abitudini da proporre e le cattive compagnie da evitare. Certamente, la Ministra ha preso le distanze: non sapeva, non poteva immaginare. Ma ha anche

Per questo, come Sinistra Italiana, abbiamo rivolto, e continuiamo a rivolgere un appello alla ministra Lorenzin: di restituire dignità al suo ruolo, di restituire dignità

Non ha bisogno di una Ministra che non ha ritenuto neanche doveroso venire a confrontarsi con l'Assemblea del Senato. Evidentemente, questo è il pieno discredito delle istituzioni portato avanti dalla Ministra e da tutto il Governo.

una cattiva comunicazione? Sì, certamente. Una comunicazione che ha messo anche in imbarazzo molte persone? Certamente sì. Ma è per questo che un Ministro deve dimettersi? Il Ministro ha posto delle problematiche molto vere ma, essendo questa un'Assemblea parlamentare dove ci sono tante anime pure che dimenticano anche la loro

spontaneamente e che questo dato è esattamente il doppio rispetto a quello di venti anni fa? É vero o non è vero che la denatalità in Italia ci vede come fanalino in Europa?

È vero o non è vero che tutte le problematiche di tipo sanitario che comportano l'infertilità non sono conosciute dal 60 per cento dei cittadini italiani?

troppo distante da ciò che possiamo capire noi; parliamo di infertilità, parliamo di fertilità, parliamo di procreazione, parliamo del desiderio dei genitori di diventare padri Parliamo di questo. E allora sulla denatalità abbiamo incombenti problematiche di crisi economica. Certo, la società italiana è profondamente cambiata È vero che le problematiche sociali sono aumentate. É vero che il problema lavorativo è drammaticamente presente nel desiderio di diventare genitori.

il ministro Lorenzin si è occupata proprio di questo problema. È vero o non è vero che la prevenzione che un tempo si faceva oggi è sconosciuta? Neanche i medici di medicina generale spesso e volentieri la fanno. Un tempo c'era il servizio militare e, almeno per i maschietti, la prevenzione dell'infertilità era presente; oggi non si fa più neanche quella. Lei, signor Sottosegretario, ha parlato dell'endometriosi e, quindi, di malattie veramente gravi. Lo sappiamo o meno che il 30 per cento di chi soffre di endometriosi è infertile? E guardate che dieci anni fa di endometriosi ne parlavano gli specialisti e questa patologia non era entrata neanche nei piani sanitari nazionali. Questo Ministro l'ha fatta rientrare nel Piano sanitario nazionale, così come si è preoccupata di affrontare

Se si vuol parlare del perché le donne non fanno figli in giovane età e si parla dell'Europa, bisogna dire che in Svezia le mamme hanno quattrocentottanta giorni pagati di congedo parentale, che possono essere distribuiti nei primi otto anni di vita del bambino. Tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro al mese per i bambini fino a diciotto anni. Per quanto riguarda la conciliazione di vita e lavoro, i giorni di permesso per restare a casa con i figli malati sono pagati e illimitati. In Francia, dal quarto mese di gravidanza, sono previsti 185 euro al mese, oltre a un premio di circa 900 euro alla nascita. Sono previsti l'allocazione familiare e 130 euro al mese fino al compimento del diciottesimo anno di età.

dovete prendere seriamente il problema della possibilità di creare una famiglia e di consentire a uomini e donne di mettere al mondo un figlio in giovane età perché hanno garanzia di poterlo mantenere, curare e farlo vivere in maniera dignitosa altrimenti il vostro Piano per la fertilità non vi dico dove ve lo potete mettere perché sinceramente è una delle cose più vergognose, sessiste e

di veder approvata una legge sugli *screening* neonatali che salvano la vita di chi fa i figli. I figli li facciamo e, quando li facciamo sani, ancora adesso non c'è la possibilità di individuare patologie curabili entro le prime quarantotto ore. È stato grazie al Movimento 5 Stelle e a una Commissione che si è spogliata dall'appartenenza politica che è stata approvata una legge perché era giusta.

donne e di natalità, si mettesse in testa che la prima cosa che una donna desidera è probabilmente avere un figlio. È naturale; è nel suo stesso essere donna

innanzitutto valuta le possibilità di consentire al figlio di vivere una vita. Questo Paese non glielo consente. Questo Governo non fa nulla per agevolare tutto questo. Pensateci bene la prossima volta. Signor Presidente, avevo preparato un intervento nel merito, ma dopo aver sentito la Capogruppo, senatrice Bianconi,

se danno garanzie. Dunque, stipulano un mutuo trentennale, dopo di che, magari, decidono di fare dei figli. Ma qual è la posizione di questo Governo e di questo Paese nel merito del sostegno alla famiglia? Non mi pare che sia la

perché le mance non risolvono il problema, servono solo a fare un po' di campagna elettorale. Poi c'è un altro aspetto da considerare: il Ministro della sanità che ha queste buone idee, secondo me avrebbe dovuto avere il coraggio di presentarsi stamattina a difendere la propria posizione, non mandare il Sottosegretario a difendere iniziative che non gli sono proprie. Questo avrebbe dovuto fare un Ministro serio. E soprattutto, mi aspetto che nella prossima legge di stabilità, al di là delle chiacchiere che vengono fatte, ci siano risorse adeguate, non campagne promozionali:

se vogliono andare in pensione per dedicarsi alla famiglia o ai figli, devono stipulare un nuovo mutuo ventennale per poter andare in pensione. Se queste sono le proposte di questo Governo e di questo Ministro, Dio ce ne scampi, perché un conto è parlare e un conto è proporre concretamente iniziative che mancano. Mi auguro che alla prossima legge di stabilità

questo Governo si rivolge all'Europa chiedendo di avere maggiore flessibilità, cioè di fare maggiori debiti da tramandare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Se questo è l'interesse per la famiglia, ripeto, sarebbe meglio cambiare registro.

il dibattito questa mattina purtroppo si è concentrato sui contenuti e sui giudizi che sono stati dati sulla campagna comunicativa del mese scorso.

credo sia necessario superare tali personalismi con equilibrio ed entrare nel merito delle politiche che possiamo individuare e promuovere per la salute riproduttiva degli uomini e delle donne.

riorientino i propri contenuti rispetto a scelte che sono fondamentali. Che cosa è importante?

di grande decadenza in questi anni perché sono stati trascurati dal livello centrale, dal livello regionale e dal livello aziendale. I consultori devono essere il luogo in cui le donne e gli uomini non si sentano lasciati soli, ma si sentano accompagnati, sia nella fase precedente

ma soprattutto dopo. Infatti, il problema è che cosa fanno le amministrazioni pubbliche nel momento in cui i bambini nascono, nei loro primi anni di vita e, soprattutto, di fronte alle enormi difficoltà che le donne incontrano nella società moderna quando hanno un figlio piccolissimo dunque un intervento specifico per sostenere i consultori e garantire una corretta applicazione della legge n. 194, che troppo spesso e sempre più frequentemente fa fatica ad essere adeguatamente sostenuta. poi un intervento attraverso le scuole. Il Sottosegretario ha parlato di politiche intersettoriali e non mi sembrava vero ascoltare questa precisazione rispetto agli orientamenti che vogliamo seguire. Politiche intersettoriali: in primo luogo, dobbiamo lavorare insieme alle scuole,

Signor Presidente, prendo la parola per fatto personale in rapporto a valutazioni di cui mi si è fatto oggetto nell'intervento del senatore Calderoli nella seduta antimeridiana del giorno 5 ottobre. Tali valutazioni sono state richiamate in Aula la mattina seguente dal senatore Centinaio. Verrò subito al punto, prescindendo dalle invettive di una volgarità da suburra indirizzatemi sorprendentemente - dopo tanti anni, davvero, non me lo aspettavo - dal Vice Presidente del Senato. E in un caso come questo si ingiuriano non un singolo, ma le istituzioni. Il senatore Centinaio ha preferito ricorrere in modo velatamente diffamatorio a espressioni derisorie per me come persona anziana. Su questi aspetti di linguaggio e costume dei due interventi non ho nulla da aggiungere. Suppongo se ne potrà parlare, nell'interesse della nostra istituzione, in sede appropriata. Il punto politico che ho ragione di considerare grave sta nell'affermazione del senatore Calderoli, richiamata in Aula la mattina seguente dal senatore Centinaio, secondo la quale io avrei «tolto a questo ramo del Parlamento la dignità definendo indegno il Parlamento». Si tratta di allusioni alla risposta che diedi a braccio alla domanda di un giovane che, il 1° ottobre al corso di formazione politica dinanzi al quale ho presentato una lezione su temi politico-istituzionali. Prima di abbandonarsi a un giudizio simile sul «collega ex Presidente della Repubblica», il senatore Calderoli avrebbe avuto il dovere di documentarsi, o almeno di attenersi a quanto le agenzie di stampa, a cominciare dall'ANSA, avevano riferito. Reagendo a forme di difesa puramente retorica del Parlamento, avevo risposto a quel giovane, denunciando - cito l'ANSA «Come si è ridotto il Parlamento» per effetto del ricorso dilagante da molti anni alla decretazione d'urgenza e a voti di fiducia su maxiemendamenti e articoli unici, che, almeno dal 2007, stravolto il processo legislativo e mortificato le Camere. E aggiungevo - cito ancora l'ANSA -: «Tutto questo può finire con la riforma costituzionale sottoposta al *referendum* per i rimedi che appresta in proposito. Questa è la sostanza: riabilitare il ruolo del Parlamento», restituendogli piena dignità. Naturalmente, sarebbe stato possibile, volendolo, documentarsi ulteriormente su quella mia breve risposta. Dire, dunque, che ho definito indegno il Senato, il Parlamento è affermazione non solo deliberatamente falsa ma opposta al senso e alle parole effettive di quel mio intervento. Da deputato per trentotto anni, da Presidente della Camera e infine da Presidente della Repubblica, ho sempre operato per valorizzare il ruolo del Parlamento e rafforzarne la funzionalità e il prestigio. Chiunque, per polemica elettorale in vista del *referendum*, tenda a negare e a macchiare questo mio incontestabile e costante comportamento, viene meno a ogni regola di minima oggettività e di rispetto istituzionale.

Signor Presidente, non sono un diffamatore di professione e non intendo offendere nessuno. Ho rispetto delle istituzioni, ma sono anche un politico e quindi, quando una persona scende in politica, anche se fa il Presidente della Repubblica ma fa politica, anche se è un ex Presidente della Repubblica ma fa politica di parte, dev'essere disponibile al confronto e, come si suol dire, a "darle" ed eventualmente a "prenderle". Non c'è bisogno di troppe citazioni per ricordare

Ha citato una *lectio magistralis*, ma si è dimenticato di citare la sede: non era la Normale di Pisa, ma la scuola di formazione politica dei Dem, che mi sembra sufficientemente di parte e politica. Riprendo quanto è stato riportato dalla stampa per poter essere altrettanto puntuale e preciso, dove si dice: «Tra decreti e fiducie, il Parlamento è stato ridotto uno straccio».

Ricordo a me stesso l'articolo 87 della Costituzione: chi autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, come i disegni di legge di conversione dei decreti-legge? I Presidenti della Repubblica. Chi promulga le leggi dopo che sono state convertite con più o meno fiducie? I Presidenti della Repubblica. Quindi, se qualcuno ha fatto girare gli stracci non è il sottoscritto ma qualcun altro che quei provvedimenti li ha firmati. Ripeto: far «votare una finanziaria con un unico articolo e 1.300 commi significa uccidere il Parlamento». Benissimo, io però ho buona memoria:

di solito l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma francamente citare episodi del genere mi sembra fuori luogo. A seguire: «Se vince il *referendum* istituzionale, avremo la possibilità di tornare a rendere il Parlamento un luogo degno». Se devo, attraverso l'approvazione di una riforma, far tornare ad essere degno, come luogo, il Parlamento, vuol dire che in questo momento è indegno per naturale conseguenza.

regolarmente eletto da parte dei cittadini, con questa congiura, è stato mandato a casa. Forse l'indegnità del Parlamento deriva dal fatto che abbiamo un Parlamento che ha espresso la fiducia a tre Presidenti del Consiglio successivi, che non sono stati mai eletti dal popolo vero, infatti, che il Presidente del Consiglio non deve ricevere il voto diretto dei cittadini, ma è anche vero che la parte che dà la maggioranza o meno all'attuale

Forse indegno è un Parlamento che ha espresso per tre volte la fiducia - e qualcuno le ha lasciate mettere - per l'approvazione della legge elettorale, cosa che è accaduta solo con la legge Acerbo e con la legge truffa. Indegno è aver fatto votare, con il ricatto dello scioglimento anticipato della legislatura, quella riforma costituzionale in cui nessuno credeva. Indegna è quella riforma costituzionale.

Indegna è la campagna elettorale e mediatica del sì, che si sta svolgendo, dove da mattina a sera vediamo solo Renzi e non c'è nessuno che faccia un minimo richiamo.

in occasione di un compleanno del presidente Napolitano. Ho detto: «Caro Presidente, auguri! Lei è come il vino rosso, come l'amarone, che migliora ad ogni anno che passa». Devo ricredermi, perché anche i migliori vini, con troppi anni, rischiano di andare in aceto.

l'indegnità del Parlamento è maturata per lungo tempo. Già il senatore Calderoli ha ricordato all'Assemblea e anche al presidente Napolitano tante cose singolari che sono accadute negli anni. Se l'interpretazione autentica del senatore e presidente Napolitano è quella che ci ha dato poc'anzi,

contestò al Parlamento di non aver approvato con la maggioranza assoluta, alla Camera, una norma sull'assestamento di bilancio da cui in quella fase, nel 2011, si trassero conseguenze mentre, l'altro giorno, presidente Grasso,

Credo che ognuno abbia diritto di esternare il proprio pensiero: il presidente Napolitano è un politico e può dire quello che vuole, ma anche noi siamo stati testimoni di storia e abbiamo assistito a tante cose indegne che sono accadute in questa Repubblica.

e la propria campagna anche sul *referendum*; tuttavia - lo dico con garbo anche al presidente Napolitano - sono stati esercitati dei ruoli, come il suo quale Presidente della Repubblica,

seria, questa sì, e molto approfondita su cosa è accaduto negli ultimi anni rispetto alla diminuzione dei poteri del Parlamento, rispetto all'uso e all'abuso dei decreti-legge.

Il problema però è che non si può dire oggi - e su questo sono molto chiara - che con questa riforma si torna

questi elementi non si possono tacere. Poi, ognuno farà la sua campagna, potrà motivare come vuole il sì e il no, ma non si può dimenticare tutto quello che è accaduto in questi due anni e il ruolo che direttamente anche il Presidente

abbiamo visto emergere una questione un po' troppo grande per un dibattito di fine seduta, mi riferisco alle prerogative del Capo dello Stato. Tra l'altro, siamo in una giornata nella quale ci accingiamo a commemorare un ex Capo dello Stato e, da questo punto di vista, se il senatore Calderoli me lo consente, con tutta l'amicizia che ho per lui, quel paragone finale enologico forse era inopportuno in una giornata come questa. Consentitemi però un'altra riflessione. Ho l'impressione che il dibattito si sia spostato su questa

sulle parole adoperate il giorno prima, in un comizio a Treviso, nei confronti di alcuni colleghi senatori,

l'aggettivo «indegno» non dobbiamo mai usarlo, neanche per fatto personale, tra di noi. In quell'occasione, a Treviso, come ha ricordato il senatore Centinaio, il Presidente del Consiglio aveva francamente adoperato termini che, se fossero stati

moderiamoci tutti, stiamo tutti attenti. Ricordo che quella mattina il presidente Zanda, anche per facilitare il fluire dei nostri lavori, riconobbe la serietà

durante i lavori della Costituente, non si occupò della Costituzione, non si sedette mai sui banchi del Governo e fu un buon esempio di discrezione.

l'amico, se ancora me lo consente, Calderoli. A parte che c'è un ordine sparso ormai, però poi il senatore Zanda avrà l'onore di concludere questa discussione. vorrei ricordare a quest'Assemblea e specialmente all'ex Presidente della Repubblica che è lui l'artefice di tutto con un intervento per fatto personale quando personalmente è entrato a gamba tesa nell'istituzione del Parlamento, quando per tre volte ha dato mandato di Governo a persone non volute Ricordo che la ministra Boschi in un'intervista ha dichiarato che il secondo mandato accettato dal Presidente della Repubblica è stato proprio in forza di questa riforma. Evitiamo allora di fare questi interventi che non servono certo a far risollevare questo Parlamento dalla decadenza in cui lo avete portato voi tutti.

sicuramente, non ha bisogno di lezioni o commenti da parte di chi, in passato, si è comportato spesso molto diversamente e non in conformità alle regole di stile che questo Parlamento merita.

ha chiesto la parola per essere stato offeso in Aula. Non ha affrontato questo aspetto dei dei nostri lavori e ha chiesto soltanto di essere interpretato per ciò che ha detto. E lo ha fatto leggendo le agenzie di stampa che riportavano con esattezza il suo pensiero. Ne è seguito un dibattito che ha affrontato il tema del funzionamento del Parlamento, che ha affrontato la questione dei poteri di firma del Presidente della Repubblica, che ha affrontato il tema della campagna elettorale, del sì e del no, dei comportamenti del Presidente del Consiglio. Ebbene, voglio dire qualcosa di generale, signor Presidente. Ci sono dei segni, degli indici, sul declino dei Parlamenti. Ci sono dei segni dai quali si può dedurre il declino dei Parlamenti. Uno di questi segni è certamente quando non si parla a tono, quando si risponde parlando di altro. Questo lo si può fare nelle conversazioni private, non si deve fare in Parlamento, dove si deve rispondere

sul profilo personale di uno di noi. È una cosa che non si fa. È una cosa che segna il declino del Parlamento. Dico invece al senatore Calderoli invece al senatore Calderoli che non si può essere Vice Presidente la mattina e senatore, con comportamenti opposti, il pomeriggio. Qualcosa che non si fa

Queste cose, senatore Calderoli, non si fanno, nemmeno nella peggiore e più violenta polemica politica. Signor Presidente, in altri tempi le parole del senatore Calderoli sarebbero state censurate. Questo non è accaduto, e anche questo è un segno del declino del Parlamento.

intervengo per fatto personale, anche se, prima di intervenire per fatto personale, ricordo che non si può essere Presidente del Consiglio la mattina*,

e magari non riesci a portare a casa la pagnotta. Presidente Zanda, lo ricordi al suo Presidente del Consiglio. Intervengo per fatto personale semplicemente perché vorrei ricordare a tutti che ho portato rispetto

in data 24 maggio 2016 affermò: «In Italia abbiamo la Lega, che è diventata la principale espressione in Italia di posizioni xenofobe». xenofobe». Penso che una persona che fa politica non possa affermare con coscienza che un partito ha posizioni xenofobe, soprattutto se è un ex Presidente della Repubblica.